è in corso la diretta televisiva della RAI. I senatori hanno facoltà di rivolgere le loro domande al Ministro per due minuti ciascuno. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, discutere oggi di politica energetica nazionale significa parlare di promozione delle energie rinnovabili, di efficienza energetica e di valutazioni sull'opportunità di riprendere in Italia la produzione di energia da fonte nucleare. Su quest'ultimo punto è da condividere la scelta del Governo di prevedere una moratoria di un anno per l'avvio delle procedure autorizzative degli impianti, al fine di approfondire tutti gli aspetti legati alla sicurezza degli impianti. Su questo anche il Parlamento farà la sua parte con l'avvio di un'apposita indagine conoscitiva, promossa dalla 10a Commissione e già autorizzata dalla Presidenza del Senato. Per quanto riguarda invece le fonti rinnovabili, prendiamo atto con soddisfazione del lavoro che il Ministero dello sviluppo economico sta svolgendo in queste settimane per giungere ad un provvedimento condiviso sul tema degli incentivi alle fonti rinnovabili. Ricordo che la Commissione industria del Senato, che mi onoro di presiedere, aveva approfondito questo tema attraverso un ciclo di audizioni di tutti i soggetti interessati, esprimendo un parere al Governo in vista del decreto legislativo adottato poi ai primi di marzo. Tra i punti qualificanti del parere, che era stato giudicato equilibrato da tutti i soggetti interessati (operatori, associazioni del settore delle rinnovabili ed istituti bancari), si era chiesto di ridurre progressivamente il sistema degli incentivi, garantendo però, al contempo, un quadro normativo certo a tutti gli investitori, soprattutto con riguardo agli investimenti già avviati o programmati. Si era infine posta l'attenzione sulla necessità di contrastare efficacemente fenomeni fraudolenti, che rischiano di danneggiare tutto il settore della *green economy*. Il Senato ha successivamente approvato in quest'Aula, con voto quasi unanime, una serie di mozioni sulle fonti rinnovabili in cui si richiamavano i principali aspetti del parere. Tali mozioni hanno sicuramente costituito un valido punto di riferimento per il Governo. Alla luce dei lavori che si stanno svolgendo presso il tavolo avviato dal Ministero dello sviluppo economico con tutti gli operatori del settore, si chiede pertanto di conoscere quali siano le decisioni che il Governo sta per assumere con riguardo agli incentivi del cosiddetto "quarto conto energia" per il settore fotovoltaico, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli investimenti già avviati; per ridurre il costo degli incentivi attualmente gravanti sulle bollette dei cittadini e delle imprese; per proseguire nell'azione di contrasto di eventuali fenomeni speculativi e fraudolenti.

ha espresso contrarietà per la scelta del ritorno all'utilizzo del nucleare per la produzione energetica. La prima argomentazione, da sempre sostenuta in quest'Aula, è la totale mancanza di credibilità economica dell'opzione nucleare, tanto più grave per l'assenza di un Piano energetico nazionale che valuti costi e benefici economici, ambientali e tecnologici e le condizioni di sicurezza delle diverse opzioni energetiche. I recenti eventi verificatisi in Giappone hanno reso impellente la definizione di adeguate garanzie per la sicurezza nucleare. In sede europea, il Consiglio dei ministri europei dell'energia, il 21 marzo scorso, ha deciso di sottoporre a *stress test* gli impianti di produzione di energia nucleare, e ciò non solo per quelli di vecchia generazione, ma anche per quelli di nuova generazione. Le autorità di sicurezza francese, finlandese e del Regno Unito, in relazione alla realizzazione di impianti EPR di ultima generazione, hanno richiesto al costruttore di dimostrare la sicurezza dei sistemi di controllo e comando del reattore. Tale vicenda interessa l'Italia, in considerazione degli accordi industriali che prevedono la costruzione nel nostro Paese di reattori EPR. Il Governo reintroduce il nucleare in Italia senza una strategia energetica nazionale, pur prevista come necessaria dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono a chiedere al Governo, che ha fissato una moratoria di un anno all'introduzione del nucleare, se non sia il caso di sospendere le procedure e l'*iter* legislativo relativo alla realizzazione di impianti nucleari; di riconsiderare gli accordi industriali sulla costruzione di reattori EPR;

Signor Presidente, onorevole Ministro, il nostro Paese ha fatto propria la direttiva UE nel campo della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, non solo condividendo l'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici, ma anche per intraprendere la strada della diversificazione nell'approvvigionamento energetico. Tra le fonti rinnovabili, quella fotovoltaica, grazie anche al sistema degli incentivi, è stata quella che più di altre si è sviluppata e si sta sviluppando al di sopra di ogni aspettativa. prova l'enorme gradimento dei cittadini nei confronti di questo tipo di energia rinnovabile, le più di 1.000 aziende che operano nel settore, i 15.000 posti di lavoro diretti ed i 100.000 indiretti, con un volume d'affari stimato dai 6 agli 8 miliardi di euro. Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2011, che blocca al 31 maggio 2011 le tariffe incentivanti, siamo vicini alla paralisi della filiera italiana del fotovoltaico

Ricordo che il 16 per cento della produzione energetica nazionale è di origine idroelettrica, e che tale percentuale è significativamente incrementabile senza ulteriori utilizzi di acqua, ma solo con l'adeguamento tecnologico attraverso il potenziamento degli impianti esistenti. L'idroelettrico interessa anzitutto i territori di montagna, contribuendo al controllo idrogeologico del territorio ed ha, quindi, una grande valenza ambientale. Il sistema degli impianti idroelettrici coinvolge interessi e partecipazioni degli enti locali, ai quali, comunque, al termine delle concessioni, ritorneranno gli impianti stessi. Qual è quindi l'orientamento del Governo verso il comparto idroelettrico in generale? Nella bozza di quello che poi è divenuto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo scorso, sul tema era previsto un riconoscimento di incentivi, rispetto ai quali le competenti Commissioni parlamentari avevano subordinato il loro parere favorevole ad una proroga di due anni. Nel testo del conseguente decreto legislativo ogni accenno esplicito all'energia idroelettrica è scomparso. Poiché gli interventi di potenziamento e rifacimento totale o parziale degli esistenti impianti idroelettrici richiedono almeno tre anni per il completamento dell'istruttoria, si pone la questione - quantomeno - delle iniziative progettuali (una dozzina in tutta Italia, mi si dice) già intraprese in questi ultimi due o tre anni, per le quali sono già state investite risorse sulla base del vecchio sistema di incentivi. Le banche, nell'incertezza del prosieguo, congelano i finanziamenti; le aziende proprietarie vivono l'incertezza per gli investimenti in cantiere. Quale è dunque l'orientamento del Governo sullo specifico delle iniziative progettuali di potenziamento e rifacimento totale o parziale degli impianti idroelettrici, attualmente *sub judice* per quanto attiene gli incentivi? Non potrebbe prevedersi, solo per tali casi, il proseguimento della pregressa modalità di incentivazione?

noi riteniamo che la ricerca e la promozione di fonti energetiche alternative rinnovabili, nonché delle tecnologie mirate alla riduzione delle fonti inquinanti rappresentino per il nostro Paese, oltre che un impegno a livello comunitario e internazionale, anche una grande sfida alla quale dobbiamo saper rispondere. Riteniamo altresì che la politica energetica sia l'asse portante di un Governo che si fa vanto quantomeno di essere un Governo del fare, che mira alla concretezza, all'innovazione, alla modernità e allo sviluppo. Senza una politica energetica considerata come asse strategico, tutti questi obiettivi non si possono raggiungere. Abbiamo registrato con positività il fatto che lei abbia comunque proposto una moratoria una moratoria del nucleare, ma riteniamo che una politica energetica seria debba avere un ampio paniere entro il quale muoversi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese, fondamentale alle nostre imprese, nonché per garantire anche tutte le tutte le dovute cautele rispetto all'ambiente, all'inquinamento e alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali. La mia domanda è imperniata su un punto fondamentale: nel nostro Paese vi è stato un arrembaggio da parte delle multinazionali straniere allorché gli altri Stati europei hanno

per regolamentare un mercato che può essere oggetto anche di interventi malavitosi e per dare certezza agli investimenti effettuati, anche in funzione del contenimento della nostra capacità di inquinare, che deve essere modulata all'interno dei parametri europei?

ripristinando gli incentivi per le fonti rinnovabili pulite e abbandonando il programma nucleare, costoso e pericoloso, su cui i cittadini voteranno il 12 e il 13 giugno per per cancellare la subdola moratoria di un anno e la mistificazione che nasconde alle autonomie locali e ai cittadini la conoscenza di come e dove si intendano costruire gli impianti.

anche riguardo al cosiddetto parco tecnologico che il Governo vorrebbe far nascere in Basilicata, con un ampliamento esagerato e sospetto del centro ENEA di Rotondella (già bocciato da un movimento popolare *bipartisan* nel 2003), che passerà da una costruzione di 6.000 metri cubi ad una di 23.000 metri cubi, con un assurdo aumento di circa il 400 per cento. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, la scelta del Governo di una moratoria sul ritorno dell'Italia alla produzione di energia nucleare è caratterizzata da una forte emotività, a seguito del disastro di Fukushima. È quindi difficile accettare che la risposta ad un tema così importante sia segnata quasi esclusivamente dall'emotività e non tenga in considerazione quanto il nucleare sia importante per lo sviluppo socio-economico dell'Italia. Ma quasi con le stesse reazioni il Governo si è posto rispetto ai numeri fuori controllo degli incentivi alle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, con un'azione che ha allarmato gli operatori perché veniva paventato il blocco totale. Infatti, di fronte ad un sistema - come accertato dal Ministero delle attività produttive - di crescita esponenziale di impianti solari e fotovoltaici, i cui oneri incentivanti si vanno a scaricare sulla bolletta con un costo di 3,5 miliardi di euro l'anno per i prossimi vent'anni, si è ritenuto di regolamentare e rimodulare il piano di incentivi. Tuttavia, le modalità di attuazione dei dispositivi correttivi, come abbiamo avuto modo di dire in altra occasione, dovranno recuperare il fatto che gli interventi autorizzati hanno un *iter* di realizzazione significativamente lungo, che l'allaccio non dipende dalle imprese, ma dall'ENEL e che il controllo del GSE è molto lento. Tale comportamento avrebbe evitato di gettare nel panico gli operatori e di dare un'immagine poco razionale delle scelte. La necessità per l'Italia, Nazione dipendente pressoché dalle forniture energetiche straniere, di avere un mercato sicuro delle forniture stesse, che per essere tale non può che essere diversificato e comprendere pertanto anche l'energia nucleare, è una condizione di sicurezza nazionale. È perciò imperativo per la nostra Nazione dotarsi di un piano energetico che abbia una temporalità di sviluppo, che preveda una molteplicità di combustibili e di modalità di produzione di energia e non sia soggetto continuamente a cambiamenti profondi sulle scelte strategiche, sovente strettamente dipendenti dal cambio dei Governi.

le domande sono molte e abbastanza complesse, alcune di carattere generale, altre particolari. Siccome non mi piace rispondere leggendo, cercherò di dare una risposta complessiva. Parto dalla senatrice Sbarbati,

nel senso che la moratoria di un anno che abbiamo immaginato per l'investimento nel campo del nucleare ci obbliga oggi, sostanzialmente, a rivedere anche il Piano energetico nazionale complessivo.

al campo energetico ed alla produzione di energia elettrica. Rimane quindi un problema complessivo da definire; probabilmente il nostro Paese ha oggi l'occasione e la necessità di rivedere le politiche energetiche nazionali.

e quindi dai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo riceviamo una fornitura molto importante. Ecco perché il Governo italiano si è mosso. Personalmente mi sono mosso con grande vigore con il commissario Oettinger che, ad esempio, intravedeva, per la strategia complessiva europea, una fornitura che partiva dall'Azerbaigian con il gasdotto Nabucco, il che non era, a nostro avviso, come Governo italiano, in linea con la strategia di distribuzione dell'approvvigionamento del

che sarebbe collegato con il *North Stream* e che tenderebbe a bypassare l'Ucraina. Nell'Ucraina oggi passa il gas russo e quindi ci sarebbe un problema di compatibilità, ma anche di contiguità e di bontà di rapporti che verrebbero

e personalmente il Ministero che dirigo, si è posto con largo anticipo nella condizione di individuare una soluzione. Sapete che in Europa la sponda Sud è sempre considerata meno importante, tant'è che il commissario Oettinger, in una sua

Devo dire che, tutto sommato, a conclusione di un lungo, e a volte anche duro, colloquio con il commissario, la sua eccentricità di interesse per il Nabucco si è molto ridimensionata. Quindi, oggi siamo in grado di competere nell'ambito delle strategie europee di approvvigionamento del gas in maniera assolutamente paritaria rispetto agli altri Paesi.

Il problema che ci siamo trovati di fronte, e che ho cercato in Commissione di descrivervi, tanto che in quella sede ho parlato sostanzialmente del peso in bolletta che ci sarebbe stato nel caso non fossimo intervenuti, ve lo ripropongo da un altro punto di vista.

Non è però possibile attivare il sistema tedesco se l'incentivo è eccessivamente alto, perché si rischierebbe di avere tanti piccoli effetti Alcoa. Ne abbiamo già avuto uno colossale, e non ne vogliamo riprodurre altri. Allora, il problema è di individuare un regime di transizione;

un monitoraggio di un livello che sia accessibile, accettabile per coloro che fanno questo mestiere, per gli italiani che hanno voglia di avere il fotovoltaico, per le aziende che hanno voglia di investire in questo settore, senza le speculazioni di cui parlavo prima, ma nel contempo attivando un percorso, un *decalage* degli incentivi che ci possa agganciare il 1° gennaio 2013 al sistema tedesco. Queste sono le cose che stiamo facendo: sono molto faticose, ma ritengo che abbiamo fatto bene a farle. È ovvio - e questo è il terzo punto - che ciò va fatto molto velocemente.

sicurezza coinvolge anche la scelta del deposito nazionale. È ovvio che questo aspetto è centrale nella nostra ricerca di obbiettivi per quanto riguarda il nucleare.

cento per rifacimento totale rispetto alla tariffa prevista per i nuovi impianti); quote annue di potenza che evitino picchi di aumento degli oneri e quindi dei prezzi dell'energia; esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e delle opere obbligatorie per legge.

penso che lo scenario e la strategia del Ministro siano convincenti, così come penso che la Conferenza nazionale sull'energia sia ormai necessaria, e quindi non più rinviabile.

Per chi ci ascolta vorrei precisare che, quando parliamo di EPR, non facciamo riferimento ad una tecnicalità particolare, ma al tipo di centrale nucleare che è previsto venga insediata in Italia, dopo che le Autorità per la sicurezza francese, finlandese e del Regno Unito

che forse il Ministro che non c'era ha sbagliato a fare i conti e che coloro che hanno fatto investimenti in questo settore si trovano adesso in una situazione di difficoltà che noi tutti conosciamo e che in Commissione abbiamo con lei condiviso. Si Si tratta di affrontare ora, con la serietà che non c'è stata prima, un argomento che è davvero vitale per il progresso delle piccole e piccolissime imprese del nostro Paese.

al sistema dei pompaggi allo studio, spero in notizie più ampie e positive, soprattutto perché alcune proposte che ho visto, ad esempio con riferimento a bacini lacustri importanti del nostro Paese, potrebbero avere dei risvolti ambientali piuttosto delicati. **Saluto

Anche questo però è un bene non rinnovabile, che quindi va assolutamente tutelato, perché fa parte dei beni paesaggistici e ambientali. Ministro, probabilmente lei era già convinto che non sarei stato soddisfatto delle sue risposte, per cui ha addirittura evitato di rispondere.

si è scelto il nucleare e si sono tagliate le sovvenzioni per le energie rinnovabili, come invece avviene in tutto il mondo; non ha risposto sul parco tecnologico della Trisaia di Rotondella. Altro che trasparenza, signor qui c'è qualcosa che non funziona e, continuando il silenzio del Governo, a titolo personale, mi rivolgerò all'autorità giudiziaria per capire quello che succede, visto che il Governo non risponde. Il reattore numero due di Fukushima ha ripreso a rilasciare liquidi e fumi, per cui l'energia nucleare non va messa nel cassetto per rispolverarla tra un anno, ma va messa direttamente in cantina. Per questo l'Italia dei Valori si appella ai cittadini, perché cassino questa avventura nucleare, e siamo convinti che il 12 e 13 giugno questo succederà.

e per l'attenzione che ha riservato alla soluzione di problemi connessi alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Mi dichiaro, pertanto, soddisfatto.